Onorevoli colleghi, è presente in tribuna un gruppo di studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Lagrangia» di Vercelli. Rivolgo a loro il cordiale saluto della nostra Assemblea. Onorevoli colleghi, ricordo che, come convenuto nella Conferenza dei Capigruppo e già preannunciato all'Assemblea martedì scorso, d'ora in poi i senatori che intendano iscriversi a parlare sull'ordine dei lavori dovranno darne previa comunicazione alla Presidenza specificando l'oggetto del proprio intervento. La Presidenza, valutata la reale attinenza delle richieste all'andamento dei lavori, si riserva di dare la parola ai richiedenti salvo casi eccezionali - a fine seduta per non più di tre minuti. Questa mattina, data la gravità della questione relativa al crollo della scuola di Rivoli e alla morte dello studente Vito Scafidi, sulla quale hanno chiesto di intervenire i senatori Ghigo e Magda Negri, sarà data loro la parola immediatamente. Ne ha facoltà. GHIGO *(PdL)*. Signora Presidente, colleghi senatori, sabato 23 novembre, alle ore 10,45 circa, si è verificato il crollo di un controsoffitto nell'aula della IV G del liceo «Darwin» di Rivoli, in Provincia di Torino. Sulla base dei primi accertamenti si sarebbe trattato di un cedimento strutturale, forse determinato dal forte colpo della porta di sicurezza di acciaio, che avrebbe sbattuto a causa del vento, provocando il cedimento dei tiranti in ferro che sostenevano la controsoffittatura. Un tubo di ghisa, caduto nel crollo, ha determinato la morte dello studente diciassettenne Vito Scafidi e il ferimento grave di un coetaneo, Andrea Macrì, attualmente ricoverato al CTO di Torino con il rischio di paralisi permanente. Il crollo ha provocato il ferimento, per fortuna in misura lieve, di altri compagni di classe, già dimessi dai presidi ospedalieri. Desidero sensibilizzare l'Assemblea su questo grave fatto, che ha profondamente scosso l'opinione pubblica non solo piemontese ma italiana, che ha portato alla morte di uno studente e ha provocato grave sconcerto per il livello di sicurezza degli istituti scolastici in tutto il Paese. il Paese. Partecipando ad una fiaccolata svoltasi a Rivoli nella serata di domenica 24 ho avuto modo di esprimere la solidarietà del Senato alle famiglie così duramente colpite dall'evento, ai compagni di scuola, ai docenti e agli amministratori locali. Ritengo opportuno che sulla vicenda e sul più complesso problema della sicurezza degli edifici scolastici, ma anche delle altre sedi (ospedali, uffici pubblici, carceri), il Senato convochi un rappresentante del Governo per riferire in merito alle iniziative da assumere e alle risorse da assegnare definendo precise priorità d'intervento.

Il procuratore Guariniello, che ha dimostrato estremo senso del dovere, precisione e coraggio, aiuterà tutti, insieme alle istituzioni, a fare chiarezza. A noi legislatori compete una scelta politica forte. Mi associo, pertanto, a quanto già affermato dal collega Ghigo che mi ha preceduto.

perché lo chiede l'opinione pubblica, lo chiede il dolore della famiglia e lo chiedono la nostra ragione, la nostra consapevolezza. Se il 40 per cento degli istituti non è a norma

determinazione, lo scavo, l'indagine, la cura del patrimonio edilizio scolastico, il coordinamento fra le istituzioni

Signora Presidente, intervengo in quanto parlamentare del territorio dove è avvenuta questa tragedia. Intendo unirmi al cordoglio, che è già stato espresso dal senatore Ghigo, anche a nome del mio Gruppo. Desidero soprattutto sottolineare che il problema della sicurezza degli edifici scolastici, come spesso capita in Italia, viene all'attenzione dell'opinione pubblica quando succedono delle tragedie.

È evidente che la responsabilità degli accadimenti nel caso di specie verrà accertata dalla magistratura, ma è importante che da oggi in avanti si pensi in modo serio a stanziare risorse ingenti, perché sappiamo che i lavori di manutenzione vengono effettuati dall'ente Provincia, che ha in capo a sé la responsabilità amministrativa

Presidente, colleghi, vorrei unirmi ai sentimenti di cordoglio e di solidarietà che sono stati portati alla famiglia

e tornano all'attenzione dell'opinione pubblica e del Parlamento. A mio avviso dobbiamo renderci conto che

ambito sociale in caso di disastri nazionali. Ritengo quindi che si debba ritornare a verificare la staticità, soprattutto, di questi istituti.

Signora Presidente, anche noi ci associamo al dolore delle famiglie di Vito e degli altri ragazzi per questa vicenda che - lo dico senza polemica - non è stata una tragica fatalità. Se delle scuole italiane deve occuparsi la Protezione civile significa che esiste un problema, che non è legato a questo o a quel Governo, bensì ad una cultura di governo locale e nazionale che ha messo gli investimenti nell'edilizia scolastica all'ultimo posto tra i suoi pensieri. Questo è il dato su cui tutti dobbiamo riflettere, dai Comuni alle Province, alle Regioni, allo Stato. A memoria, l'ultimo piano straordinario importante di investimenti nell'edilizia scolastica risale ai tempi della ministro Falcucci. Da allora tanta acqua è passata sotto i ponti; le competenze dei Comuni e delle Province in tema di edilizia scolastica sono aumentate, le risorse a disposizione di questi enti si sono progressivamente ridotte e sono anche vincolate ai limiti del patto di stabilità previsto per le autonomie locali. Questo modo di concepire il sistema delle priorità e dei bisogni dei cittadini da tutelare è anche causa di queste tragedie

una scuola degna di un Paese civile e non sudamericano, con tutto il rispetto per il Sud America.

ringrazio, senatore Di Giovan Paolo. La sua richiesta sarà fatta presente ai Capigruppo e alla Giunta per il Regolamento proprio per ottemperare in tal senso; andremo in quella direzione.

il decreto-legge in esame, nella prospettiva di rilanciare la competitività del settore agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale, reca taluni interventi relativi all'adeguamento della normativa agricola nazionale alla disciplina comunitaria, al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo, alle agevolazioni fiscali nel settore delle bioenergie, alcune disposizioni relative agli enti irrigui, come pure la soluzione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per gli anni 1994-1999. Il decreto-legge si rende necessario ed urgente in quanto detta disposizioni in grado di rimediare alla situazione di debolezza strutturale del comparto,

ad un impiego efficace ed efficiente delle risorse destinate all'amministrazione dell'agricoltura. Nella fattispecie si evidenzia che l'articolo 1 del decreto-legge n. 171 del 2008 modifica la disciplina del credito d'imposta, così come definita dall'articolo 1, commi 1088, 1089 e 1090 della legge n. 296 del 2006. La modifica si è resa necessaria in quanto solamente nel febbraio del 2008 la Commissione europea ha approvato lo schema del decreto attuativo degli aiuti previsti dalla legge n. Va ricordato, infatti, che la legge finanziaria per il 2007 è entrata in vigore il 1° gennaio 2007, mentre lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di attuazione della legge n. 296 del 2006, è stato predisposto e diffuso nel luglio del 2007. La modifica in questione riconosce ad alcune categorie di imprese di beneficiare del credito d'imposta sino al 50 per cento delle spese ammissibili, escludendo altresì dal beneficio di cui trattasi le imprese agroalimentari di grandi dimensioni, fatta eccezione per il regime *de minimis*. Pertanto, il provvedimento va accolto con favore dal momento che risponde alle esigenze delle imprese che intendono crescere sui mercati esteri ampliando le proprie quote di mercato. Inoltre, lo strumento è senz'altro innovativo e può contribuire ad aumentare significativamente la propensione all'*export* nell'agroalimentare italiano. Rispetto al testo della legge finanziaria per il 2007, va valutato positivamente il fatto che le percentuali del valore degli investimenti, escluse dalla base imponibile del reddito d'impresa, siano state unificate ad una sola (per il 50 per cento), mentre precedentemente risultavano diversificate e 50 per cento, a seconda dei casi). Va, peraltro, rilevato un aspetto "politico" del provvedimento, vale a dire che i beneficiari della misura possono avvalersi del «credito d'imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo», «purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa»: tale vincolo deriva dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Passando all'esame degli articoli, la lettera *a)* dell'articolo 1 del decreto-legge in esame novella il comma 1088 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconosce, per il biennio 2008-2009, alle imprese che realizzano prodotti di cui allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché a favore delle piccole e medie imprese - come definite dal regolamento n. 70/2001 della Commissione,

anche alle imprese non rientranti nelle categorie indicate alla lettera *a)*, sia pure nei limiti del regolamento comunitario sugli aiuti di importanza minore. La lettera *c)* modifica parzialmente il testo del comma 1090 della legge finanziaria per il 2007. In particolare, quest'ultimo estendeva il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, anche se con un'attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. La predetta lettera *c)* elimina il riferimento al lavoro autonomo, contenuto nel vecchio testo del comma 1090. Viene inoltre soppresso il terzo periodo del comma 1090, che nel testo originario attribuiva agli imprenditori agricoli, in alternativa alla esclusione della base imponibile, il beneficio del credito di imposta, per un ammontare pari ad un terzo di quello previsto nei commi 1088 L'articolo 2 disciplina l'assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato. Si segnala a tale proposito che nell'anno 2007, in base a quanto previsto dai commi 2 e 2*-bis* dell'articolo 22*-bis* del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il contingente di 250.000 tonnellate annue di biodiesel fiscalmente agevolato è stato suddiviso in una quota prioritaria

viene previsto che tale beneficio venga attuato prioritariamente a favore del biodiesel da filiera, tramite i criteri fissati da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi del comma 1 del citato

non è allo stato attuale ancora avvenuta. Dal punto di vista finanziario, come precisato anche nella relazione illustrativa, l'articolo 2 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) di prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e la distribuzione dell'acqua. La gestione commissariale non è stata, peraltro, in grado di far fronte agli impegni finanziari, sia per la deficitaria situazione di bilancio, sia per le azioni esecutive promosse nei confronti della stessa, che non consentono atti dispositivi del patrimonio. Per far fronte a tale situazione il decreto-legge in esame, all'articolo 3, comma 1, attribuisce all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) un contributo straordinario di 5.600.000 euro per far fronte agli impegni derivanti dalla gestione ordinaria fino al 31 dicembre 2008. Il comma 2 del predetto articolo 3, in considerazione dell'eccezionale esposizione debitoria e al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di distribuzione dell'acqua, stabilisce che le somme erogate non siano soggette ad esecuzione forzata per un periodo limitato e, particolarmente, fino al 31 marzo 2009. Il comma 3 dispone che, per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, l'organo esecutivo dell'EPLI destina le somme erogate esclusivamente alla gestione ordinaria. Il comma 4 proroga di un ulteriore anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano, istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048, che cesserebbe la propria attività il 7 novembre 2008, 2008, qualora non si intervenisse con un nuovo provvedimento di proroga. L'attività istituzionale dell'ente, a seguito del trasferimento di alcune competenze alle Regioni, avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica n. 616, si è sviluppata essenzialmente nel campo della progettazione e della realizzazione, nelle aree territoriali delle Regioni Umbria e Marche, di grandi opere idroelettriche di accumulo e adduzione delle risorse idriche e nella gestione delle opere stesse per scopi irrigui e civili, in base alle concessioni di derivazioni di cui è titolare. L'articolo 4, nella prospettiva di risolvere un'emergenza di carattere finanziario e gestionale correlata ai tempi e alle procedure contabili nazionali ed europee (relativamente, in particolare, agli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura orientamento della pesca (SFOP)), porta a conclusione il pregresso amministrativo-finanziario della programmazione per gli anni 1994-1999, ponendo i relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro, a carico del Fondo di rotazione, di cui del 1987, istituito nell'ambito del Ministero del tesoro. Peraltro, questa conclusione positiva eviterà il blocco degli interventi dello Strumento finanziario di orientamento alla pesca per gli anni 2000-2006, sempre a cofinanziamento europeo ed in scadenza entro la fine del corrente anno. In conclusione, signora

dove mancano all'appello diverse risorse sia per quanto riguarda l'anno 2008, sia per quanto concerne la programmazione dell'anno 2009. Sappiamo che per l'anno 2009 mancano all'appello 230 milioni di euro

Altri argomenti su cui si è discusso sono l'interpretazione autentica in materia di ICI (cioè sulla ruralità dei fabbricati a disposizione degli utenti agricoli)

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il decreto in esame contiene misure che di per sé condividiamo, perché interventi nati nella scorsa legislatura attendevano un completamento con l'adeguamento alle normative comunitarie per diventare operativi e permettere agli imprenditori del settore di usufruire di agevolazioni entro il 2008. Così è per la misura che riguarda il credito di imposta per la promozione e i provvedimenti per la pesca. Così, urgente è l'assegnazione del biodiesel defiscalizzato perché gli operatori possano programmare i contingenti assegnati. Con senso di responsabilità non ci opponiamo alle proroghe e ai contributi straordinari che riguardano gli enti irrigui, perché sappiamo essere a rischio i servizi idropotabili, pur avendo in merito opinioni diverse e ravvisando l'urgenza di un intervento più strutturale. Nel merito delle singole misure, dunque, non possiamo essere contrari e ne ravvisiamo certo il carattere d'urgenza, tanto che noi stessi abbiamo proposto emendamenti per inserire nel decreto provvedimenti che riguardano la tenuta del settore della pesca in grande difficoltà, le agevolazioni previdenziali che riguardano le zone montane e le zone svantaggiate, il Fondo di solidarietà per gli incentivi assicurativi (i cui mancati rifinanziamenti stanno mettendo in ginocchio migliaia di imprenditori) e altri che riguardano incentivi attraverso crediti d'imposta, imprenditoria giovanile e femminile, trovando su alcuni emendamenti anche convergenze su soluzioni minimali con la maggioranza. Questo per dire di un atteggiamento di grande senso di responsabilità che il nostro Gruppo sta assumendo: abbiamo tenuto in Commissione e lo teniamo in Aula cercando di capire quale sarà la risposta del Governo e se ci saranno altrettanta consapevolezza ed altrettanta responsabilità. Diciamo con forza che non c'è proporzione tra ciò che il settore in questo momento sta vivendo e l'esigua, inadeguata risposta che questo Governo sta dando: l'inadeguatezza dello strumento e dei provvedimenti che il Governo utilizza per affrontare la crisi di un settore agroalimentare - che sta vivendo una delle fasi più critiche che abbia mai conosciuto. Lo hanno detto nei giorni scorsi migliaia di imprenditori, di operatori del settore, che sono andati in piazza e non per voglia di movimentismo gratuito, ma perché i segnali che arrivano dal mondo agricolo sono allarmanti. La difficoltà è reale. I numeri sono allarmanti. Sono oltre 200.000 le imprese agricole a rischio chiusura, oltre il 10

C'è un livello diffusissimo di indebitamento delle aziende così come non si era mai visto prima, non per investire ma per gestire l'esistente. I redditi sono in caduta libera ed il calo è il più marcato tra i Paesi europei. Diverse aziende stanno producendo in perdita. in perdita. Signora Presidente, nella zona da cui provengo, una delle più ricche del Paese, la zona del parmigiano reggiano, solo nella mia Provincia, Reggio Emilia, sono 120 le aziende che chiuderanno il 31 dicembre. Mai visto prima! Non riesco ad immaginare cosa può succedere nelle zone più deboli. Le cause sono diverse e purtroppo concomitanti. È l'impennata dei costi di produzione (ovvero energia, carburante, materie prime, mangime nella zootecnia, costo del lavoro, degli oneri sociali e delle assicurazioni). È la difficoltà di accesso al credito, appesantita dalla crisi finanziaria, con la contemporanea difficoltà degli istituti di credito. A tutto ciò vanno aggiunte le condizioni internazionali completamente modificate, che evidenziamo come una crisi congiunturale diventa a questo punto crisi strutturale profonda nel settore. È un vero e proprio cambio epocale cui stiamo assistendo e a cui le nostre aziende non possono far fronte da sole. Per decenni il reddito dell'azienda agricola si è formato in dipendenza di tre fattori: un mercato molto regolato; politiche di sostegno alle produzioni; tutela dei prodotti nel loro ingresso sul mercato. Oggi lo scenario è completamente cambiato, oggi si viaggia in mare aperto. L'accordo dei giorni scorsi a Bruxelles ha sancito definitivamente la chiusura di un'epoca e l'avvio di un'altra, che parla di liberalizzazioni, mercato e, insieme, di garanzia di qualità del prodotto e di qualità ambientale. Ci sono passaggi del tutto inediti. Lo stesso incremento immediato delle quote latte sarà un elemento che, da un lato, se non troverà un sistema solido a gestirlo, potrà diventare ulteriore fattore di fluttuazione del prezzo del latte e dei suoi derivati dall'altro, se verrà confermato il contenuto del verbale sottoscritto dal nostro Ministro a Bruxelles, potrà essere una deriva e comportare un rischio di accettazione dell'illegalità. Ci auguriamo ancora che non sia così. Dico questo perché credo che la politica debba comprendere quanto sia grande e inedita tale fase. Siamo passati dalla formazione del reddito in agricoltura in un contesto di garanzie senza rischio di impresa a un tempo, quello attuale, in cui l'azienda opera in un contesto di fortissima competizione internazionale e, per contro, in una realtà nazionale caratterizzata da un preoccupante calo dei consumi. Di più, le dinamiche dei mercati, la centralità della questione alimentare, le strette correlazioni tra qualità dei prodotti e qualità ambientale e la destinazione a fini energetici dei prodotti agricoli hanno cambiato la natura stessa della professione dell'agricoltore. Si è passati da un produttore agricolo a cui era chiesto, come dice la parola, solo di produrre ad un imprenditore agroalimentare ambientale che deve conoscere i mercati, creare valore con nuove strategie e con un riposizionamento della propria azienda, tutelare l'ambiente, ricercare, innovarsi ed utilizzare nuove tecnologie. A nessun altro comparto credo venga assegnata tanta responsabilità. Ad una sfida di questa portata non si risponde solo con misure tampone, tampone, ma con una proposta strutturata, con politiche organiche, con una finanziaria che metta al centro la questione alimentare, capace di traghettare il settore e diventare sistema; misure che incentivino aggregazioni delle imprese per affrontare con determinazione la sfida dell'internazionalizzazione (perché lì ci sono i nuovi mercati), che incentivino fortemente la crescita di una nuova imprenditorialità, il ricambio generazionale e l'imprenditoria femminile (perché lì c'è la possibilità di futuro). Ma, prima ancora, la condizione preliminare è la garanzia di un quadro di stabilità, perché solo in esso può nascere un'imprenditoria vera. Non si chiedono garanzie assistenzialiste, ma stabilità sì. Per quanto riguarda la previdenza, occorre rendere stabili e strutturali gli interventi agevolativi sulla contribuzione previdenziale. Occorre poi rendere stabile il sistema di protezione dai rischi che, per chi produce alla mercé delle influenze climatiche, diventa decisivo. Occorre rendere stabile il sistema fiscale, che va misurato sulle caratteristiche del settore e sulle sue peculiarità e non considerato come sistema di risulta Lo diciamo qui oggi, lo abbiamo detto e lo diremo in finanziaria: questo dovrebbe essere l'approccio di responsabilità serio che un Governo dovrebbe adottare verso il secondo comparto economico del Paese.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il provvedimento in esame, che reca misure urgenti per il rilancio competitivo del comparto agroalimentare, come diceva la senatrice Pignedoli, è stato valutato positivamente dal mio Gruppo in Commissione

Come sottolineava la senatrice Pignedoli, il Partito Democratico vuole contribuire con responsabilità per scongiurare la crisi del comparto agroalimentare e vuole mettere a disposizione del Governo le proprie proposte. Lo stesso testo del decreto ha infatti visto impegnato il Gruppo del Partito Democratico in proposte emendative, raccogliendo anche i giusti appelli che in questi giorni ci sono venuti dalla Confederazione italiana agricoltori e dalla Confagricoltura, che condividiamo pienamente e che meriterebbero risposte adeguate come la predisposizione di un pacchetto di misure per favorire gli investimenti e per sostenere un settore fondamentale, quello agricolo, che è a rischio di recessione, come è emerso anche dalla recente ricerca ISTAT sullo stato di salute dell'agricoltura italiana. italiana. Il Partito Democratico fin dall'inizio della legislatura ha richiamato l'attenzione del Governo e della sua maggioranza sull'esigenza di prevedere investimenti adeguati a sostegno del comparto agricolo, piuttosto che tagli su importanti voci di spesa che avrebbero messo gravemente a rischio il settore. Si deve constatare che nei primi mesi del Governo i provvedimenti adottati a sostegno del rilancio competitivo di un settore che sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua recente storia sono stati parziali e inadeguati a fornire risposte efficaci agli agricoltori italiani. La dimostrazione è stata l'assenza di una strategia politica sul settore agroalimentare all'interno tanto del DPEF quanto del decreto‑legge n. 112, in cui non hanno trovato collocazione interventi per lo sviluppo del comparto, né tanto meno sono stati previsti stanziamenti. La stessa finanziaria per il 2009, pur contenendo alcune misure per il comparto agricolo e della pesca, richieste a gran voce in questi mesi proprio dai senatori del Partito Democratico in Commissione agricoltura, non garantisce gli interventi necessari per il consolidamento e lo sviluppo del nostro sistema agroalimentare.

fare alcun investimento di rilievo in un settore che per competere ha bisogno invece di innovazione e di ricerca, di crescita dimensionale, di sostegno alle imprese colpite da calamità e da crisi di mercato. È necessario, quindi, che il Governo riveda la propria posizione e sia disponibile ad accogliere gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico per affrontare le questioni più urgenti e reperire le risorse per finanziare il Fondo di solidarietà nazionale per il triennio 2009-2011, al fine di dare piena attuazione ai meccanismi di gestione del rischio in agricoltura e potenziare il ruolo delle polizze Riteniamo questo uno strumento di vitale importanza per arginare i rischi che contraddistinguono l'attività agricola, riteniamo urgente intervenire per il rifinanziamento del piano irriguo nazionale al fine di favorire l'avvio e il completamento delle opere in esso previste e fronteggiare e superare le situazioni di emergenza idrica che colpiscono soprattutto le Regioni del Sud. Questa emergenza la sta vivendo in questo momento la nostra Regione, la Basilicata, che, insieme alla regione Puglia, ha chiesto e ancora non ottenuto dal Governo il riconoscimento dello stato di crisi. Riteniamo poi fondamentale estendere il credito d'imposta a tutto il territorio nazionale, confermare le agevolazioni in materia previdenziale per il triennio 2009‑2011 nelle aree montane

sviluppare interventi che siano volti a ridurre la lunghezza della filiera agroalimentare. Occorre inoltre prevedere un piano specifico di interventi a favore del settore cerealicolo, anche per contrastare le tante speculazioni che producono le impennate dei prezzi dei prodotti a largo consumo, come pane e pasta, e sostenere il settore dell'olivicoltura. Credo sia necessario, anche rispetto al momento che sta vivendo il comparto agroalimentare, favorire l'accesso al credito e la ristrutturazione finanziaria delle nostre imprese. imprese. Vorrei concludere dicendo che, a mio avviso, attraverso l'adozione di queste misure da parte del Parlamento potremo trarre l'agricoltura fuori dalla marginalità in cui è stata relegata e reinserire il settore sul sentiero dello sviluppo e della competitività. *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi senatori, onorevoli rappresentanti del Governo, la complessiva difficoltà che ha investito l'economia del Paese mette a nudo la situazione di debolezza strutturale dell'intero comparto agricolo, un settore primario, protagonista nella produzione di beni alimentari di prima necessità. Assegnare all'agricoltura quel ruolo e quella funzione strategica nei prossimi anni diventa oggi obiettivo irrinunciabile. Ritengo fosse questa l'intenzione del Governo quando ha varato il decreto-legge n. 171, nella consapevolezza, o meglio, con il proposito di mettere in vigore da subito, data la straordinarietà del momento, misure urgenti che consentissero il rilancio competitivo del settore agroalimentare italiano. Di fronte ad una situazione di difficoltà straordinaria e all'emergenza il mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare si è posto in attesa di risposte forti, convincenti, rassicuranti. Forse le attese riposte travalicano le possibilità concrete della disponibilità finanziaria, ma è altrettanto vero che ad uno ad uno stato evidente di emergenza, di crisi sul fronte dei prezzi, dei costi di produzione aumentati a dismisura, della contrazione dei consumi ci vuole una risposta coraggiosa e straordinaria. Non sono affatto convinto che il provvedimento oggi all'esame sia esaustivo per conferire quel rilancio al settore. Lo svuotamento del fondo di solidarietà nazionale viene rimpinguato solo con uno stanziamento assolutamente insufficiente a garantire i rischi sulle calamità naturali. Il piano nazionale irriguo, strumento di riferimento delle politiche mirate al risparmio idrico e alla corretta gestione delle acque, viene abbandonato spero solo rimandato a momenti successivi - ma rinunciando così alla prosecuzione di interventi, in linea con una visione moderna delle pratiche agricole e dei consumi di risorse, quelle idriche, non sempre e continuativamente disponibili. Tutti convengono che il tema della modernizzazione dell'agricoltura non può prescindere della necessità di un ricambio generazionale. Ebbene, nulla al riguardo viene esplicitato nelle intenzioni contenute nel disegno di legge in discussione, nonostante interventi emendativi ne invocassero una rinnovata attenzione verso l'imprenditoria giovanile e femminile, in grado di conferire vigore e slancio ad un settore che denuncia un tasso di età media non coerente con quella prospettiva di modernizzazione, anche anagrafica. Siamo concordi con alcune linee impostate nel provvedimento; tuttavia dichiariamo una non soddisfazione per l'inadeguatezza del pacchetto di interventi, che non trova profilo strutturato ad una domanda, anzi ad una attesa, che rimane tuttora inappagata.

momento di riflessione sull'agricoltura per porre all'attenzione alcune questioni a noi, alla maggioranza e a tutto questo ramo del Parlamento, riguardo all'incidenza del ruolo politico di questo settore a alle possibilità che abbiamo rispetto all'Unione europea. Dico questo in dipendenza innanzitutto - ci tengo a dirlo pubblicamente - della costruttività del lavoro fatto. Questo è merito soprattutto, per quanto riguarda questo ramo del Parlamento,

lo svolgimento tra maggioranza e opposizione di un confronto oggettivamente costruttivo (e il sottosegretario Buonfiglio lo ha riconosciuto pubblicamente anche nelle riunioni che ci sono state). Entrando nel merito di queste questioni, utilizziamo questo momento nel nostro ramo del Parlamento,

È stato giustamente fatto notare dal Presidente della nostra Commissione e, in particolare, dal collega Vallardi, che segue molto queste tematiche, il successo ottenuto dal Governo nelle trattative a Bruxelles. Quel giorno mi sono anche astenuto dall'intervenire perché non credevo fosse necessario distogliere l'attenzione solo perché noi siamo l'opposizione. Il nostro Paese è in ballo quando ci sono trattative a Bruxelles ed un uso migliore dei fondi

europea. Su questo ho trovato non solo legittimo, ma anche positivo - se volete - l'entusiasmo con cui il Presidente e il collega Vallardi hanno salutato questo risultato. Non staremo a sminuirlo per il fatto che sul tabacco è andata meno bene che sulla questione delle quote latte.

significa anche porci responsabilmente il problema degli altri settori. Sappiamo bene, infatti, che il tema delle quote latte è stato un problema non solamente di legalità (che va fatta crescere anche in questo mondo, ovviamente dopo trattative fatte in trattative fatte in maniera anche coraggiosa), ma anche un problema rispetto ad altre quote, perché è evidente che noi abbiamo avuto di più avendo di meno da altre parti. Questa trattativa è di tutta l'Italia. Noi allora dobbiamo sostenere il Paese e dobbiamo sostenere il sistema che noi rappresentiamo anche quando siamo in condizioni diverse di maggioranza o opposizione o di Governo. La seconda questione inerente l'Unione europea riguarda il contributo che l'Italia può dare affinché l'Unione faccia una politica moderna.

del giorno futuro.

la forza di dare all'agricoltura un ruolo anche nel futuro dell'Europa e non solamente per la conservazione e la difesa di ciò che abbiamo. Questo è un compito che dobbiamo svolgere assieme, perché significa mettere in gioco le nostre relazioni con i consumatori, ossia le relazioni con la vera cittadinanza europea del futuro.

delle norme di legalità e un modo di vivere nella logica della legalità che potrebbe cancellare tutte le sanzioni e le infrazioni su cui abbiamo avuto difficoltà. Ritengo

può mettere il nostro settore in grado di risultare determinante nella conservazione del territorio, nel rapporto con i poteri locali e - mi rivolgo ai colleghi della Lega - con un federalismo vero, radicato all'interno del territorio. Vi è la possibilità di costruire qualcosa di più ampio, ossia un rapporto tra il Nord e il Sud del mondo più equilibrato, fondato su un regime di natura, che non è il diritto naturale, ma ciò che assieme, come esseri umani, abbiamo costruito in questi anni.

Sulla scia del collega Di Giovan Paolo, intendo prendere a pretesto i temi che il nostro relatore, senatore Piccioni, ha così brillantemente illustrato, per allargare il discorso (anzi, il cono d'ombra che vorrei eliminare con un fascio di luce più ampio e potente) a tutto il comparto agricolo, del quale credo di interpretare i sentimenti, soprattutto di coloro che vi si muovono all'interno e di cui forse troppo poco si parla anche in quest'Aula. Dobbiamo in effetti alla tenacia del relatore Piccioni all'appoggio fondamentale del presidente della Commissione, senatore Scarpa Bonazza Buora, se il dibattito odierno può allargarsi ad una visione che non è soltanto quella dei temi enunciati, ma riguarda anche la promozione del sistema agroalimentare all'estero, il contingente del biodiesel defiscalizzato, il funzionamento e il sostegno agli enti irrigui e la pesca, che viene sempre accomunata, con un binomio talvolta un po' bizzarro, al comparto dell'agricoltura, per quanto concerne

alle difficoltà e ai problemi che il mondo agricolo sta affrontando nell'ambito della crisi generale. Gli agricoltori, come sempre fanno, stanno affrontando difficoltà forse più grandi rispetto a quelle lamentate da settori produttivi diversi, con la dignità e la consapevolezza, che hanno sempre avuto, che debbono prima di tutto rimboccarsi loro le maniche e poi andare a chiedere aiuti altrove. proposito, il discorso sull'Europa, che il collega Di Giovan Paolo ha introdotto, è più che pertinente. Sappiamo che l'agricoltura sta andando incontro a un toboga, a uno scivolo che non ha più freni, a quanto pare, nella considerazione del bilancio comunitario.

Ed ogni volta è l'agricoltura che paga con un'erosione sistematica di questa fetta di bilancio. Eppure, guardando all'agricoltura senza fare pura demagogia, possiamo ben dire che, se andasse davvero in crisi, se dovesse profondamente non rispondere più alle istanze del mercato globale, sarebbe un problema per tutti. L'agricoltura, infatti, è un settore sinergico con molti altri. È il motore, per esempio, dell'industria agroalimentare di cui stiamo parlando, della filiera commerciale (quanti commercianti debbono ai prodotti dell'agricoltura, alla puntualità e alla loro qualità le loro fortune economiche), dei trasporti

Ma il riflesso finale, ciò che realmente dà l'idea dell'importanza e della buona salute del comparto agricolo è il mondo dei consumatori, il bilancio familiare di cui tanto oggi si discute e sul quale tante lacrime vengono versate. I consumatori sono i primi

la sfida per la qualità e i prezzi equi si vince non ostacolando soltanto la produzione degli altri, ma potenziando la produzione interna, sia europea, sia nazionale, e per potenziarla occorre aver fiducia nei vari comparti.

puntando sulla qualità. Sembra un discorso perfino banale, tanto è semplice e abusato: è la qualità che fa la differenza, oggi, nella scelta del consumatore. Ebbene, a tale riguardo sarà allora utile ricordare che l'Italia è ricca di prodotti di qualità,

formulare un suggerimento: spendiamo un po' di soldi - mi rivolgo al Governo - per aumentare i controlli su questi prodotti, per difendere la loro tipicità, spesso la loro unicità. questo caso attenzione, però, perché quando nasce un taroccamento generalmente segue un nuovo regolamento, che non solo non riesce magari a frenare chi più abilmente tarocca ancora, ma impone nuovi lacci e nuovi lacci e lacciuoli proprio a colui che all'inizio, magari in maniera spontanea, aveva iniziato a produrre qualcosa di migliore e di diverso. Quindi, auspico più incentivi a chi garantisce questa produzione di nicchia, meno regolamenti, ma anche più controlli per chi cerca di taroccare. In questo campo, vorrei invitare anche il Governo a unire, allo sforzo del settore agricolo, quello delle politiche comunitarie. Sappiamo tutti benissimo che all'ombra dei grandi edifici che ospitano le istituzioni europee, per esempio a Bruxelles, vi sono vi sono supermercati nei quali si battono record mondiali di prodotti italiani taroccati: dal prosciutto al formaggio alla pasta, qualsiasi cosa che abbia un titolo italiano viene venduto a un prezzo superiore, in confezioni direi direi smaccatamente fasulle, falsificate, eppure non vi è un controllo adeguato per smascherare queste forme di frode, di frode, non solo alimentare e settoriale, ma soprattutto comunitaria. Pertanto, alle iniziative di cui oggi stiamo parlando, vorrei unire un invito ad accelerare ed accentuare questo tipo di controlli. Infine, vorrei fare una notazione che riguarda l'insieme dei temi Abbiamo sentito anche dalla collega Pignedoli un'esortazione a capire che stiamo parlando di misure in parte iniziate dal Governo precedente (secondo noi migliorate con l'intervento attuale, ma sicuramente da condividere) che hanno una caratteristica comune: l'estrema urgenza postaci dall'Unione europea nell'applicazione di regolamenti che altrimenti verrebbero a scadere alla fine di quest'anno con grave perdita anche di risorse comunitarie.

per dare una mano agli agricoltori, che non hanno tempo di fare sciopero, signor Sottosegretario, in quanto gli animali devono mangiare tutti i giorni e quando c'è bisogno di acqua non ho mai visto un contadino che per protesta non apre un rubinetto per l'irrigazione. le azioni in campo agricolo generalmente non fanno rumore, ma scavano sempre solchi profondi. Buon lavoro.

ha richiamato l'attenzione della maggioranza sull'esigenza di prevedere investimenti adeguati a sostegno del comparto agricolo, piuttosto che tagli su importanti voci di bilancio (circa 223 milioni di euro relativi alle missioni di spesa dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze) che avrebbero messo gravemente a rischio il settore. durante il dibattito sul Documento di programmazione economico-finanziaria, in quanto membri del Gruppo del Partito Democratico in seno alla 9a Commissione, avevamo già evidenziato, i miei colleghi ed io, un'assoluta inadeguatezza rispetto alla complessità e all'urgenza delle problematiche relative a comparti delicati ed abbisognevoli di considerazione e di sostegno, come l'agricoltura, l'industria agroalimentare, la pesca e i settori connessi. Oggi, in quest'Aula, desideriamo ribadire la necessità di un'inversione di rotta da parte del Governo, di una politica di maggiori investimenti nel comparto e di provvedimenti straordinari mirati al sostegno del settore primario. In piena coerenza con l'azione che, come Partito Democratico e come Gruppi di opposizione, alla Camera e al Senato abbiamo finora portato avanti, purtroppo spesso inascoltati,

per la verità, devo dire che in Commissione, come hanno già evidenziato alcuni colleghi (per primo lo ha fatto il relatore Piccioni), abbiamo trovato massima apertura ed ascolto, condivisione e convergenza. Il presidente Scarpa Bonazza Buora ha registrato e costruito un clima di piena collaborazione di cui gli do atto e il sottosegretario Buonfiglio ha potuto assumere, nelle circostanze in cui nei giorni passati è stato presente all'illustrazione degli emendamenti, elementi sufficienti per poter riferire in merito al Governo. Il Governo, quindi, non può o non potrebbe ignorare le legittime aspettative delle categorie professionali, delle forze sociali soprattutto ora: è un dato inconfutabile che l'agricoltura sta attraversando una fase di recessione in un quadro globale gravemente colpito da una economia stagnante. I fatti ne danno dimostrazione: le manifestazioni di questi giorni, su iniziativa di di Confagricoltura e di CIA a Bologna e qui a Roma come in tutta Italia, hanno mobilitato tanti e tanti operatori del settore e testimoniano un malessere diffuso, che non può essere sottovalutato. Chiediamo al Governo e alla sua maggioranza l'inserimento di 200 milioni di euro per il Fondo di solidarietà nazionale, l'estensione del credito di imposta e dei contratti di filiera nel settore agroalimentare a tutto il territorio nazionale, il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta, la promozione della produzione di energia elettrica da biomasse, agevolazioni sulla contribuzione per le aree svantaggiate, la risoluzione dei contenziosi contributivi giacenti presso l'INPS. La senatrice capogruppo in Commissione del Partito Democratico, si è già lungamente soffermata su queste questioni ed ha anche riferito in ordine alla necessità, condivisa dal senatore relatore Piccioni, dell'avvio e del completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale. incentivazioni per l'occupazione giovanile e per la imprenditorialità femminile, aiuti concreti per i settori della pesca e dell'acquacoltura, in particolar modo l'aggiornamento della figura dell'imprenditore ittico, l'istituzione di un fondo per lo sviluppo della filiera ittica per garantire il riposizionamento e la ristrutturazione delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, ed anche l'esenzione dalla formazione del reddito dei premi ottenuti dal FEP (Fondo europeo per la pesca), l'estensione di accordi di filiera simili a quelli già previsti per il settore agricolo, la soppressione del registro delle imprese di pesca e l'esenzione dell'imposta di bollo così come stabilita per il settore agricolo. È necessario dunque mettere in campo un'azione energica e l'opportunità è data dalla conversione in legge del decreto che oggi occupa l'attenzione di questa Assemblea. Ciò, anche utilizzando qualche spunto - come ho detto in in Commissione - oggettivamente positivo contenuto nel disegno di legge predisposto dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, in modo da trasfonderlo in uno strumento più veloce, dunqueimmediatamente in grado di assicurare risposte tempestive almeno ad alcune delle istanze maggiormente avvertite dalle categorie interessate, che non possono più attendere i tempi della politica.

da una disattenzione del Governo o da un fine di non ricevere: sarebbe un peccato sciupare un impegno che la Commissione intera, senza differenze politiche, ha profuso anche fino a queste ultime ore, prima dell'inizio del lavoro in Aula, tenendo dinanzi a sé presente unicamente gli interessi alti dell'agricoltura italiana. Prima dell'approvazione della legge finanziaria il Governo può e deve dare prova della sua reale volontà di rilancio del settore e dei differenti comparti che vi afferiscono. È necessario, con l'approvazione del testo di legge e dei suoi emendamenti, dare il via ad una nuova fase di sviluppo delle qualità tipiche dell'agricoltura italiana e delle sue peculiarità, per renderla sempre più competitiva nello scenario globale.

Signora Presidente, sono costretto a dissentire con la massima energia dalla decisione, che mi si dice sia stata presa nella Capigruppo, di rinviare alla fine dei lavori dell'Aula gli interventi - pur brevissimi, e confinati in tre minuti - sull'ordine dei lavori. Devo dissentire, innanzitutto, per un motivo di ordine logico. Se si interviene sull'ordine dei lavori, si presume che si debba intervenire all'inizio:

perchè ci si trova impossibilitati a sollevare anche il problema che solo il singolo parlamentare può avere la libertà di pensare. Siamo qui tutti uguali e uno può pensare che c'è un argomento fondamentale da portare all'attenzione dei colleghi e deve avere la libertà di poterlo fare.

che dovrebbe essere chiamata correttamente Commissione per la vigilanza dei sistemi radiotelevisivi, perché, anche se si dà per scontato che non potrà mai vigilare su Mediaset, dovrebbe vigilare su tutti i sistemi radiotelevisivi. Io stesso mi ero ripromesso di intervenire su questo tema e sul fatto che si tratta ormai di una Commissione fantasma, ombra, che si riunisce a piacere di un Presidente,

di fronte a tutti i colleghi su questo argomento, ma non ho potuto farlo. Mi riprometto di presentare una memoria scritta per illustrare con la massima precisione possibile, a termini di Regolamento, tutta la questione, che considero un'ingiustizia assoluta.

Signora Presidente, desidero ricordare in maniera personale il collega Sandro Curzi, giornalista della RAI, Radiotelevisione italiana, scomparso nell'ultimo fine settimana. Desidero farlo perché appartiene a quella categoria di giornalisti e di professionisti che sicuramente ha lasciato un segno, sul quale potremo discutere a lungo, ma che innegabilmente ha dato una svolta alla qualità dell'informazione radiotelevisiva;

Eravamo abituati a muoverci all'interno di un apparato radiotelevisivo - quindi informazione pubblica - connotato da una diffusa e nebulosa presenza di partiti e di politiche, che sapevamo essere condizionanti per le carriere di tutti i giornalisti, o quasi, e dei massimi dirigenti: mai,

nei discorsi che ho sentito in questi giorni, lo hanno sufficientemente approfondito. Certamente con questa sua proposta Curzi ha tolto al giornalista radiotelevisivo quel tipo di aureola che aveva di equidistanza ed indipendenza, ma finalmente ha fatto chiarezza. Oggi forse anche alcuni suoi discepoli, titolari di rubriche prestigiose e di grande presa sul pubblico, dovrebbero ricordare questa lezione: essere di parte non può significare essere mascherati, ma coerentemente se stessi, pur in un tentativo di equilibrio. *(Applausi dei

che le nostre sedute dovrebbero essere dedicate principalmente a trattare gli argomenti previsti all'ordine del giorno e non ad una sorta di «varie ed eventuali», specialmente ad inizio seduta.

tragico fatto verificatosi nel liceo di Rivoli. Il senatore Ghigo è intervenuto a nome del Gruppo del Popolo della Libertà. Egli era sul posto la sera in cui sono avvenuti i fatti (io ci sono stato nel pomeriggio con il ministro Gelmini) e ha espresso quello che si doveva esprimere: una solidarietà alle famiglie colpite e un intendimento di lavorare per migliorare la sicurezza degli edifici scolastici; si è limitato a questo. Purtroppo gli interventi che sono seguiti hanno cominciato a parlare di responsabilità del Governo, dei tagli che hanno danneggiato questo settore, della mancanza di attenzione. Avrei voluto anche citare nello specifico quanto è stato detto,

prossimo. Se una cosa è stata ben chiara negli interventi del Governo e se vi è stata una priorità individuata con sicurezza, non dopo quello che è successo a Rivoli ma ampiamente prima, è stata proprio la questione della sicurezza degli edifici scolastici. Inviterei quindi ad evitare questo tipo di

per un fatto che non ha nulla a che fare con questi tagli, proprio i rappresentanti dei partiti che siedono nella Giunta della Provincia di Torino. Sia il presidente Berlusconi, Sia il presidente Berlusconi, sia la presidente della Regione Piemonte Bresso hanno parlato di fatalità. Se qualcuno però insiste nel cercare responsabili politici, essi non stanno certo da questa parte del Parlamento, del Parlamento, ma proprio in quella che ha voluto fare un discorso politico su una vicenda tragica che ci deve far riflettere e spingere al massimo impegno a tutti livelli.

senatore Malan con estrema lealtà - bisognerebbe ricordare l'espressione del presidente Ciampi ai funerali di quei ragazzi, il 3 novembre 2002, quando disse

Spesso, è stato detto anche in quest'Aula, dopo le disgrazie si piange e si arriva sui luoghi della disgrazia in pompa magna, ma poi questo Stato assassino dimentica le tragedie per poter operare con leggi, regolamenti e interventi vari.

Noi, nel nostro Comune, abbiamo la scuola più sicura d'Europa perché costruita sui famosi molloni sperimentali, inaugurata tanto tempo fa.

sperando fosse in un ambiente sicuro. Lo hanno affidato allo Stato, alla scuola. Tutti insieme dobbiamo lavorare stabilendo delle priorità. Il Governo precedente, caro Malan, nel 2002-2003

non solo alla mamma che ha perso il figlio ma a tutta la comunità di Rivoli, colpita da questa tragedia.

che non perde occasione per criticare l'operato di questa Presidenza. Ricordo che all'unanimità tutti i Capigruppo hanno deciso, per regolare meglio i lavori dell'Aula e per permettere all'Assemblea di lavorare, di inserire gli interventi sull'ordine dei lavori a fine seduta. Questo ragionamento è stato fatto anche con un collegamento diretto al Regolamento del Senato.

ma non usate l'Aula semplicemente per criticare a vuoto l'operato della Presidenza.

intendo aggiungere il mio cordoglio per il gravissimo incidente occorso a Rivoli, di cui alcuni colleghi hanno già parlato stamani. Penso però che sia opportuno che l'Assemblea, quando si interviene su simili argomenti, oltre ad evitare facili strumentalizzazioni politiche,

vi è stato un drammatico incidente dove abbiamo perso la vita di un giovane ed immediatamente trarre come conseguenza la mancanza di fondi è, a mio modo di vedere, un atteggiamento un po' superficiale. che in questi ultimi dieci anni la Provincia di Torino ha stanziato ben 626 milioni di euro in manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delle scuole medie superiori, delle quali è responsabile. Si tratta di circa 1.200 miliardi di vecchie lire. Come loro comprendono, si tratta di una cifra importante. Diventa quindi, a mio modo di vedere, un po' superficiale trarre immediatamente le conclusioni di una mancanza di risorse. È evidente che in questo campo le risorse non sono mai

Dobbiamo quindi ragionevolmente pensare che quanto avvenuto può essere riconducibile o ad una fatalità, come hanno detto il presidente della Provincia Mercedes Bresso e il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, o ad un errore nei sistemi di controllo e monitoraggio, o a una cattiva esecuzione dei lavori e quindi ad un successivo carente carente momento di verifica di quei lavori. Dobbiamo attendere l'esito delle indagini della magistratura per arrivare ad una conclusione, ma credo opportuno in questo momento evitare strumentalizzazioni politiche:

che siamo di fronte a un problema che non è dovuto semplicemente, come è stato detto da troppi in modo superficiale, ad una carenza di risorse, ma è probabilmente riconducibile a qualcos'altro e sarà la magistratura a verificare di che si tratta.